che, almeno in questa sede, stante l'argomento di questa settimana, mi sia data una risposta o, meglio, sia data una risposta a tutti i colleghi. In questa interrogazione chiedevo se chiedevo se il Ministro dell'economia e delle finanze non ravvisasse un conflitto di interessi nella figura del presidente e amministratore delegato della società che gestisce gli studi di settore. In effetti, il commercialista Gianpietro Brunello è amministratore e appunto, come dicevo prima, presidente di questa società che, ricordo

Nella figura di questo commercialista, che, da una parte, gestisce la società per gli studi di settore e, dall'altra, applica gli studi di settore nella sua attività di commercialista, io ravviso chiaramente un conflitto di interessi. Se il Governo potesse magari darci un cenno su questa mia

alcune questioni alla Presidenza in maniera che vi sia tutto il tempo per poterle affrontare. Esse riguardano sostanzialmente l'ordine dei nostri lavori e questo mi pare pertanto il momento più opportuno per segnalarle. Presidente, come lei sa, la Presidenza dell'Assemblea ha assunto come criterio per l'iscrizione all'ordine del giorno e per le votazioni l'ordine cronologico della presentazione delle mozioni e degli ordini del giorno.

secondo l'ordine cronologico, salvo le parti assorbite o quelle precluse. Questa impostazione, Presidente, non è proprio quella prevista dal Regolamento: quest'ultimo prevederebbe un'attivazione da parte della Presidenza

questione, Presidente, impone un chiarimento da parte della Giunta per il Regolamento. Poiché ormai accade con una certa frequenza che al momento del voto delle mozioni e degli ordini del giorno vi sia una qualche incomprensione - come è successo ultimamente proprio sulla questione Visco-Speciale - sarebbe il caso che la Giunta per il Regolamento affrontasse la materia

il criterio definitivo sul quale la Giunta per il Regolamento conviene, noi avremmo la necessità, per trasparenza di comportamenti, di sapere qual è il momento a partire dal quale sarà possibile il deposito della mozione o degli ordini del giorno e la sede

per la quale chiedo a lei di interporre buoni uffici affinché anche su di essa la Giunta per il Regolamento si pronunci. Tale questione è più strettamente relativa al merito. lei potrà constatare già sulla questione che è al nostro esame, vi sono mozioni che, in alcune parti, presentano addirittura parole simili se non uguali. Si ricorderà tutta la discussione fatta dal Presidente dell'Assemblea sulla questione dell'apprezzamento dell'operato della Guardia di finanza, ciò che ne scaturì e le discussioni che vi sono state (a dire il vero, anche le incomprensioni e gli equivoci). Signor Presidente, una cosa

ogni senatore debba esattamente sapere che cosa sta votando. Non è infatti possibile un voto su una previsione generica; si vota una determinata mozione salvo le parti precluse e quelle assorbite.

potrebbero perfino essere simili nelle parole, e comunque simili nei contenuti, che però, inserite in un contesto anziché in un altro, hanno un valore e un significato politico completamente diverso.

in relazione a quel caso, apprezzamento sull'operato della Guardia di finanza, l'altro che non era riferito al caso Visco-Speciale, ma esprimeva in generale e e in assoluto un giudizio sul ruolo della Guardia di finanza. Eppure è nata un'incomprensione: la Presidenza ha deciso che fossero la stessa cosa, noi abbiamo accettato tale decisione, ma insomma ci sarebbe stato molto da discutere. signor Presidente, sulla questione riguardante i contenuti delle preclusioni e degli assorbimenti io penso che, se vogliamo evitare alla Presidenza di turno di trovarsi

nel senso che quando i titolari o il titolare di uno strumento, sia esso mozione o ordine del giorno, ritengono che una determinata espressione, ancorché ripresa in altri documenti presentati, vada valutata nel contesto proprio dello strumento presentato, essa non può essere ritenuta d'ufficio preclusa o assorbita. Ciò perché il proponente o i proponenti ritengono

Giunta per il Regolamento in maniera che, nel prosieguo dei nostri lavori, si possa procedere con chiarezza e trasparenza e ognuno possa svolgere il proprio ruolo di maggioranza e di opposizione, e di opposizione, e anche la Presidenza possa decidere senza sollevare quei dubbi e quelle perplessità - ricordo un suo intervento proprio nell'ultima occasione - che mettono poi la stessa Presidenza in una condizione di difficoltà. rendere tutto chiaro e trasparente, penso sia arrivato il momento di un pronunciamento della Giunta per il Regolamento. Signor Presidente, la ringrazio e mi scuso se sono stato un po' lungo.

rispetto al mettere ai voti per prima la mozione su cui il Governo esprime un parere favorevole: questo è previsto per le risoluzioni sul DPEF. C'è la possibilità da parte del Governo di arrivare a questo ponendo la questione di fiducia su una delle mozioni, e quindi scegliendone una sola e solo quella. Sui contenuti, gli Uffici sono già al lavoro per verificare anticipatamente

sulla base di un'iniziativa parlamentare che non lascia dubbi quanto ad ordine cronologico di presentazione delle mozioni. Infatti, proprio al fine di ottenere la fissazione in tempi certi di questa seduta,

sull'ordine da assegnare alle mozioni (ferma restando, come lei ha bene osservato, che solo nel caso di apposizione del voto di fiducia da parte del Governo su una mozione si debba rispettare, per l'iniziativa parlamentare e i tempi e i modi con cui questa si determina), in questo caso non vi è dubbio che l'ordine di votazione debba essere quello già predisposto.

che si era manifestamente avviato nel corso del periodo precedente all'entrata in attività di questo Governo, come ha testimoniato l'andamento delle entrate nel corso del 2006, il quale si è rivelato molto superiore a ciò che ragionevolmente può attribuirsi all'andamento dell'economia, alla crescita del prodotto interno lordo. Il rispetto dei diritti del contribuente, che pure viene ricorrentemente richiamato nella mozione della maggioranza, in realtà, è stato più volte violato da questo Governo, nel momento in cui ha previsto norme che consentono all'Amministrazione finanziaria di assumere informazioni all'insaputa del contribuente, senza che questi abbia la possibilità di instaurare, rispetto all'eventuale incompletezza od erroneità di quelle informazioni, un adeguato contraddittorio.

riguardato l'ammortamento dei beni strumentali di impresa o anche a quelle di cui ora ci accingiamo a discutere. Ancora, la leale collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti non si determina, non si sollecita, non si promuove ogni qual volta l'amministrazione in senso più ampio viene meno alla parola data, e certamente la parola data anche il 16 dicembre 2006 alle 2006 alle associazioni rappresentative delle categorie del lavoro autonomo era stata nel senso della conferma di quanto già la legge istitutiva degli studi di settore disponeva nel lontano 1996: la regola per cui devono essere definiti attraverso la consultazione e la ricerca dell'intesa con le associazioni di categoria, oltre che il passaggio presso la commissione degli esperti che deve esprimere un motivato parere. Tutto ciò non è accaduto accaduto quando, il 10 marzo 2007, il Governo ha varato nuovi indicatori di normalità con i seguenti vizi fondamentali: in primo luogo, senza il parere della commissione degli esperti, né tanto meno il confronto con le associazioni rappresentative delle categorie interessate agli studi di settore; in secondo luogo, gli indicatori sono stati calibrati grossolanamente su 200 studi di settore e non sui singoli *cluster* o gruppi omogenei di imprese che sono previsti all'interno degli stessi studi di settore; in terzo luogo (e questa è la ragione più grave che determina rottura nel rapporto tra amministrazione e contribuente), questi indicatori di normalità, come elementi di ausilio ai contribuenti, nel momento cioè in cui rappresentano un *warning*, un segnale di avviso relativo al possibile accertamento che potrebbe conseguire dallo scostamento tra alcuni elementi della dichiarazione e questi indicatori di normalità, invece di un utilizzo a fini di individuazione delle attività di semplice accertamento, questi indicatori di normalità, unilateralmente e con effetto retroattivo, vengono incorporati nei meccanismi di calcolo degli studi di settore, alzano la base di calcolo e quindi le soglie degli studi di settore, con la conseguenza di legge per cui si rovescia l'onere della prova con effetto retroattivo, si determina in capo ai contribuenti una presunzione, forse anche legale, di colpevolezza, che pone in capo al contribuente l'onere della prova contraria. Il tema, quindi, è essenzialmente questo e per tale motivo la nostra mozione ha un dispositivo assolutamente semplice e chiaro: la non retroattività di studi di settore che sono stati determinati

che sono stati cioè prodotti unilateralmente secondo una tecnicalità che non ha precedenti e che non è stata oggetto d'esame né dalla commissione degli esperti, né dalle associazioni di categoria. la retroattività non dovrebbe aversi nel momento in cui non si tratta né di norma di interpretazione autentica, né di norma meramente procedimentale, perché solo ora il legislatore, in base alla in base alla legge n. 296 del 2006, ha dato questo effetto giuridico a questi indicatori e quindi allo scostamento dagli studi di settore, con la conseguenza che ho prima ricordato dell'inversione dell'onere della prova. prova. Le ipotesi che altri hanno avanzato e che avanzeranno in quest'Aula, contenute nella mozione della maggioranza, non risolvono in nulla e per nulla il problema che abbiamo sollevato, perché affermare che questi studi sono sperimentali, che questi indicatori sono sperimentali non attenua in nulla e per nulla la loro efficacia rispetto ai redditi del 2006. credo che la sperimentalità sia ovviamente in *re* *ipsa* nel momento in cui sappiamo essere già stati convocati i tavoli per la revisione periodica degli studi di settore stessi. Ma nondimeno non risolve in nulla e per nulla il problema l'ipotesi di utilizzare gli studi di settore per liste selettive di controllo, perché si tratterebbe ancora di liste ancorate alla logica dell'inversione dell'onere della prova, cioè liste selettive di controllo relative allo scostamento dagli studi di settore. Quindi, insisto con la conseguenza dell'inversione dell'onere della prova. prova. Non possiamo certo chiedere ai contribuenti di sperare che, nel periodo che intercorre tra la loro dichiarazione e il possibile accertamento, intervengano studi di settore più favorevoli. Tale è il pasticcio che il Governo ha combinato che vari sono stati i tentativi in questi giorni di porvi rimedio, ma senza mai fare quel passo indietro che noi chiediamo al Governo, quella rinuncia all'odiosa retroattività che è prevista nella disposizione. Si è pensato addirittura ad una possibilità di conguaglio a novembre senza oneri, cioè prevedendo una doppia dichiarazione dei redditi. Vedo che il buonsenso ha poi fatto sparire questa stupida

nel momento in cui il Governo si appresta ad incrementare per una entità che può andare dagli 8 ai 10 miliardi di euro aggiuntivi di spesa corrente, il Governo, ancor più in questo contesto, ha l'esigenza di incrementare la pressione fiscale già odiosamente elevata, quella stessa pressione fiscale che ha prodotto quell'odioso tesoretto che in realtà è solo il frutto di una rapina fiscale. Voi pensate cioè di ottenere un ulteriore extragettito attraverso la semplice minaccia di soglie di reddito determinate dagli studi di settore così come modificati dagli indicatori di normalità, ipotizzando che i più si adeguino pagando una sorta di pizzo istituzionalizzato per comprare la protezione dell'Amministrazione finanziaria anche se i contribuenti pensano di non dovere queste maggiori somme all'erario; voi pensate cioèche vi sia un effetto di deterrenza su coloro che già pagano le tasse, su coloro che già sono attori di un leale rapporto di collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Per noi non ci sono mediazioni, perché vi è una sola soluzione possibile per ripristinare i diritti del contribuente, ed è quella di rinunciare all'effetto retroattivo per l'anno 2006 di questi indicatori di normalità e dell'effetto che essi producono sulla base di calcolo degli studi di settore e, conseguentemente, sull'inversione dell'onere della prova che determinano. Questa e non altra può essere la soluzione che può venire dall'Assemblea se si vuole ricostruire il rapporto tra fisco e contribuente, se non si vuole che si determini quella rottura del patto sociale che nel patto fiscale ha un elemento così determinante. Per queste ragioni, sosterremo con convinzione la nostra mozione.

Per la prima volta, dopo molti anni, i dati di finanza pubblica per il 2006 sono risultati migliori delle previsioni e segnalano una tendenza assai confortante in direzione del controllo della spesa ed il risanamento dei conti;

di rivedere in crescita, con una stima intorno al 2 per cento, anche le previsioni riferite al 2007. Su questo quadro, nettamente più positivo rispetto solo ad un anno fa, hanno agito certo anche fattori esterni e di trascinamento - noi siamo a rimorchio della crescita europea e della Germania - ma non si può negare che vi abbiano avuto un peso anche le misure adottate, già a luglio 2006 e poi con la finanziaria 2007, da parte del Governo. In particolare, insieme al controllo selettivo della spesa, anche attraverso gli accordi con le Regioni per il controllo della spesa sanitaria e le innovazioni nei trasferimenti agli enti locali, nonché attraverso il sostegno ed il rilancio della spesa pubblica per investimenti, un significativo apporto alla manovra è venuto dall'impegno di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, a sottolineare una linea di intervento che si differenzia - le parole del senatore Sacconi hanno consentito di apprezzarne anche la diversità

su questo terreno è necessario costruire un grande patto, un impegno comune tra lo Stato e la platea ampia dei contribuenti leali (famiglie, lavoratori, imprese), perché è dal recupero dell'imponibile evaso che possono venire le risorse per ridurre il carico fiscale che grava su di loro e per sostenere politiche sociali e di sviluppo. L'aumento dal lato delle entrate da gettito tributario è risultato, nel 2006, assai rilevante. Questo dato di forte incremento è coerente con una tendenza registrata in molti Paesi europei. Ciò probabilmente avviene come riflesso, abbastanza generalizzato, di una serie di fattori connessi alla ripresa, che ho richiamato prima: un forte recupero dei profitti societari; un buon recupero delle componenti della domanda interna con forti ricadute sul gettito, vale a dire la spesa per i consumi; una *performance* positiva dei mercati azionari e, in alcune realtà, prezzi delle abitazioni ancora in crescita. Pur considerando questa molteplicità di ragioni a effetto diffuso, resta il fatto che una parte delle maggiori entrate sia ascrivibile, come si è opportunamente evidenziato da parte del Governo, al miglioramento spontaneo della *tax compliance* e ad altri fattori legati all'emersione della base imponibile. Si tratta di un primo confortante riscontro, posto che il contrasto all'evasione fiscale è uno degli impegni cardine dell'azione per il risanamento dei conti, il sostegno alla crescita, gli obiettivi di equità. A distanza di un anno e scontando qualche semplificazione, di cui chiedo scusa, si possono enucleare dall'insieme degli interventi attuati tre tipologie di azioni abbastanza caratterizzate nel campo degli interventi in materia fiscale. Un primo gruppo di interventi ha avuto la finalità di ampliare l'insieme delle informazioni da mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto attraverso l'utilizzo delle strumentazioni e delle tecnologie informatiche: penso all'anagrafe dei rapporti tra operatori finanziari e clienti, all'utilizzo di sistemi di tracciabilità e di moneta elettronica, all'acquisizione di informazioni già disponibili presso enti ed amministrazioni pubbliche a fini di approfondimenti e di verifiche. Un secondo insieme di provvedimenti è esplicitamente finalizzato a rafforzare la potestà e l'attività di controllo, di accertamento e di sanzione da parte dell'Amministrazione finanziaria. mi piace richiamare anche il prezioso lavoro svolto in Commissione finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento con un importante parere espresso sull'atto di indirizzo che orienta le attività dell'Amministrazione finanziaria e delle agenzie, cioè un vero e proprio *check-up* di monitoraggio sul nuovo funzionamento e sugli interventi che possono rendere più efficace l'azione e l'iniziativa di questi uffici e di queste strutture. Un terzo gruppo di interventi è volto a prevenire o contrastare specifiche attività finalizzate all'evasione fiscale. È in questo insieme di interventi che si iscrive anche l'affinamento del più importante strumento di accertamento dei ricavi dei lavoratori autonomi e delle imprese, specie di piccole dimensioni: gli studi di settore, appunto, ciò di cui discutiamo e che è alla origine delle mozioni che oggi si confrontano in quest'Aula. Gli studi di settore - voglio sottolinearlo e ribadirlo - sono strumenti statistici costruiti sulla base dei diversi fattori economici che riguardano l'attività di alcune categorie di lavoratori autonomi e di professionisti.

applicative conseguenti alla *minimum tax* e per offrire un punto di riferimento da un lato ai contribuenti, dall'altro all'amministrazione fiscale. È importante questo profilo di strumento, non contro qualcuno, ma utile a entrambi: l'amministrazione fiscale e i contribuenti. Gli stessi studi della SOSE, la società che ha il compito di predisporli, sono formulati per statuto insieme alle organizzazioni di categoria e agli ordini professionali. Questi strumenti per loro natura devono essere però sempre affinati *in progress*, sulla scorta dell'evoluzione dell'economia e delle dinamiche dei vari settori, nonché dei maggiori dati che arricchiscono le le banche di riferimento conoscitive degli enti e dei soggetti che le devono utilizzare. Richiedono quindi un periodico aggiornamento e verifiche ricorrenti di congruità.

Si è previsto che gli studi vengano aggiornati ogni tre, invece che ogni quattro anni, e si sono messi a punto nuovi indicatori di coerenza, quegli indici di normalità economica come specificati poi nel decreto ministeriale del 20 marzo 2007. L'assunto è in sé corretto perché la predisposizione di più accurati indicatori può favorire una più penetrante azione di controllo. In questo spirito, il 14 dicembre scorso, le organizzazioni rappresentative delle piccole imprese dell'artigianato, del commercio e dei servizi, hanno sottoscritto

È stato un importante risultato. In questo quadro di positiva concertazione e responsabilizzazione che ha già avviato per il 2007 la revisione di 65 studi, con la partecipazione delle categorie interessate e con l'obiettivo di determinare indicatori di normalità economica specifici e propri, si è inserita, generando grande preoccupazione e reazioni di giustificata contrarietà, un'iniziativa dell'Agenzia delle entrate che con circolari, oltretutto tardive, del 22 maggio e del 13 giugno, ha dettato disposizioni circa l'adozione degli indici di coerenza e di normalità economica, senza che fosse in merito intervenuto il confronto e l'intesa con le associazioni d'impresa e dei professionisti interessati. Non è stata certo un'iniziativa felice: voglio dirlo con molta nettezza. Il senso della mozione che presentiamo come maggioranza è dunque quello di contribuire a riportare chiarezza e serenità nel rapporto tra l'amministrazione fiscale e i contribuenti interessati dall'applicazione degli studi di settore e far sì che possa da subito ripartire il tavolo della concertazione tra amministrazioni e categorie, offrendo riferimenti certi e motivati alla platea dei contribuenti. Del resto, è positivo che il Governo abbia già confermato che l'obiettivo che si vuole raggiungere con gli indicatori di normalità economica è solo quello di contrastare taluni comportamenti fraudolenti, colpendo sostanzialmente la concorrenza sleale verso le imprese sane. Inoltre, ha aggiunto che per i controlli sulle dichiarazioni del 2007, che saranno effettuati a partire dalla fine del 2008, si applicheranno, se più favorevoli ai contribuenti, gli studi revisionati e, ancora, che queste innovazioni sono sperimentali per consentire al contribuente che non si sia adeguato in dichiarazione di poter chiedere - come recita anche il riferimento nel testo della mozione - nell'eventuale contraddittorio dell'accertamento con adesione, l'applicazione dello studio a lui più favorevole tra quello del 2006 e quello a regime. Infine, si è definito il posticipo del pagamento delle imposte al 9 luglio senza maggiorazioni, in modo da consentire ai contribuenti e agli intermediari fiscali di conoscere e valutare meglio tutta la problematica in questione. Prendendo positivamente atto - come dicevo - di tutto questo, la mozione della maggioranza rende però esplicita e rafforza una serie di indicazioni che, che, confermando la validità delle linee della politica fiscale del Governo, vuole contribuire ad avviare, dopo lo sforzo di risanamento di questo primo anno, una fase di positiva collaborazione, aprendo una fase nuova di maggiore corresponsabilizzazione nel campo dell'attuazione delle politiche per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Questo a partire proprio dal riferimento agli obiettivi che sono richiamati nella mozione del DPEF, laddove si prevedeva, in un quadro coerente di più generali azioni per il *welfare* e il sostegno alle fasce deboli della popolazione, di destinare le maggiori entrate derivanti dalla lotta alla evasione fiscale, permanenti ed eccedenti gli obiettivi di risanamento, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale. Questo impegno va ribadito con forza perché i buoni risultati di risanamento e sostegno alla crescita sono però temperati da un livello della pressione fiscale che è al 42,3 per cento del PIL, un dato che si conferma anche con lieve incremento per il 2007 e che richiede dunque - come noi auspichiamo - che già per il 2008, nel DPEF in preparazione, sia ragionevole attendersi l'individuazione di un obiettivo di pressione fiscale discendente in modo graduale per i prossimi anni. Inoltre, la mozione sottolinea l'importanza che si operi per migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria e che il sistema fiscale sia improntato al riconoscimento del primato dei diritti del cittadino contribuente, fondato su regole più semplici e certe - la semplificazione è una esigenza indifferibile ormai - e con aliquote più adeguate e proporzionate. In particolare, con riferimento agli studi di settore, si raccomanda - le nostre sono indicazioni puntuali, pertinenti ed utili a dare esecutività efficace, certa e positiva anche alle esigenze rappresentate dalle categorie - di interpretare come sperimentale la disposizione recata nell'articolo 1 della legge finanziaria, sottolineando che l'introduzione degli indicatori di normalità economica deve avvenire con l'ausilio irrinunciabile delle associazioni di categoria interessate, restituendo questi studi e questi indicatori alla funzione originaria - come evidenziato nel protocollo del 14 dicembre - cioè di segnali di anomalia meritevoli di approfondimento; i segnali di anomalia meritevoli di approfondimento vanno seguiti e ottimizzati, perché servono a fare una seria lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. fiscale. Poi, proprio per questo, quegli indicatori di normalità economica, data la loro natura sperimentale, devono essere utilizzati proprio al fine della costruzione delle liste selettive di controllo, senza nessun automatismo accertativo. Questo mi pare sia il nucleo fondante della nostra indicazione operativa per superare la situazione di incomprensione e di difficoltà, oltre che il metodo della concertazione da riprendere che accompagna l'impianto della mozione. Infine, si sottolinea anche l'esigenza di prevedere nel testo della mozione l'emanazione di ulteriori istruzioni applicative, che auspichiamo siano rapide e sollecite dopo questa discussione, a seconda di come essa si concluderà, per individuare criteri oggettivi al fine di identificare meglio le situazioni di marginalità economica, per le quali non si rendono applicabili gli indicatori stessi, e che siano poi emanate direttive per una forte azione di informazione e formazione volta a migliorare il contraddittorio tra i contribuenti e gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate. Non possiamo ignorare che in materia di studi di settore va rafforzata la cultura della consulenza e della collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, utile a favorire un dialogo fecondo, costruttivo, efficace e soddisfacente per il contribuente stesso. Più in generale - e mi avvio a concludere, signor Presidente -, la mozione di maggioranza coglie anche l'occasione per sollecitare il Governo, allargando l'ambito dell'attenzione, a valutare la possibilità che sia rivista la disciplina relativa all'obbligo di presentazione dell'elenco clienti-fornitori, nel senso di esonerare da questo adempimento, per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, almeno per alcune tipologie di importi e di volume di attività. Infine, a fissare la scadenza per l'invio telematico del modello Unico al 30 settembre 2007, stanti le numerose novità e gli aggravi di adempimenti introdotti dalla recente normativa e dalle circolari applicative emanate

al 30 settembre è quanto mai auspicabile. Infine - lo diciamo spesso ma vorremmo fosse davvero assunto nella sua pregnanza e forte rilevanza di indirizzo di indirizzo - auspichiamo si faccia ogni sforzo per migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria attraverso uno scrupoloso rispetto dello Statuto del contribuente, rafforzando gli strumenti di consultazione preventiva con le associazioni di categoria e le organizzazioni rappresentative degli intermediari fiscali. Con queste indicazioni, signor Presidente, come maggioranza siamo fiduciosi - sostenendo con convinzione gli obiettivi del Governo di politica fiscale e di lotta all'evasione e all'elusione - che questi indirizzi, se tradotti appropriatamente, possano risultare utili a rendere più incisiva l'azione dell'amministrazione fiscale nel perseguimento dei suoi obiettivi di interesse generale: ciò proprio in ragione del supporto che a questi obiettivi e a questa azione può venire da una maggiore comprensione e condivisione degli stessi obiettivi da parte dell'opinione pubblica e delle diverse categorie dei contribuenti. *(Applausi

è aumentata la pressione fiscale (siamo oltre il 42 per cento); è aumentato il debito pubblico italiano; la spesa pubblica è aumentata di 8 punti

Probabilmente tutte le politiche adottate dal Governo in materia economico-fiscale sono state sbilanciate: un dato che a noi preme continuamente evidenziare è che si continua a dimenticare la struttura portante dell'economia italiana.

L'ossatura di questo microsistema imprenditoriale produce l'85 per cento del prodotto interno lordo. Perché solo i piccolissimi riescono ad avere questi risultati? Innanzitutto, riescono ad avere una grandissima elasticità gestionale; sopravvivono a tutte le crisi momentanee di medio termine perché non fanno altro che aumentare il tempo che dedicano all'attività,

un grande debito: esse vivono esclusivamente grazie ai sostegni pubblici che, di volta in volta, vengono sistematicamente erogati. Se verifichiamo dove sono finite le grandi imprese italiane viene da mettersi le mani nei capelli! La grande distribuzione è sostanzialmente in mano ai francesi. Delle due ultime grandi banche, Antonveneta è finita sotto controllo olandese;

dell'Alitalia, ma è probabile che finisca sotto il controllo russo. Signori, Governo o chi lo rappresenta in questo momento, vi state rendendo conto che ci resta solo questo microsistema di imprese, che continuate a vessare in modo

Ma è possibile ideare un sistema che pone fuori della normalità il 70 per cento delle piccole imprese?

È meglio nazionalizzare tutto: faccia tutto il Governo; assuma queste microimprese e stabilisca come devono operare e che tipo di reddito lasciare all'operatore che, a questo punto, diventerebbe un subordinato.

non sono 3 lire! La media di aumento per ogni impresa si aggira tra i 9 ed i 10.000 euro. Ciò sta a significare che l'imposta da pagare per ogni impresa rispetto all'anno precedente sarà di 3.000 euro. Precedentemente avevamo già il 30 per cento delle imprese

che valuta, con parametri probabilmente molto efficaci, l'intensità dell'evasione fiscale Regione per Regione.

di fare dei sacrifici per trascinare vagoni che, dai dati economici dei Ministeri, risultano inesistenti sotto il profilo economico? Non credo che in Calabria si viva peggio che in Emilia, in Veneto

Sulla base di quali accertamenti? Sulla base numerica di quante valutazioni e verifiche aziendali? Chiudiamo questo capitolo, ma è indubbio che c'è anche un aspetto geografico, di non poco

Il reato economico sembra essere la peggiore infamia, la peggior cosa, il pericolo sociale più alto da dover combattere con tutti i mezzi. È strano vedere come si tollerino tutte le devianze, tutti i malcostumi, l'uso di droga, persino la disubbidienza e i reati comuni; si preferisce fare un indulto piuttosto che un condono fiscale,

sul lavoro irregolare il cui aspetto peggiore è la criminalizzazione del datore di lavoro che sbaglia, nell'assumere: è meglio che vadano a fare i criminali piuttosto che dare un lavoro al limite della legalità.

sarà di 0,50 euro; per questa somma lo Stato preferisce chiudere un'attività (da tre giorni in avanti) e rinunciare a tutto l'introito. Questo ci fa capire quanto masochismo c'è in chi pretende un rigore sotto il profilo economico che non ha ragion d'essere, a questi livelli. Adesso stiamo attenti - questo è un monito rivolto al Governo - perché avete tanto pestato piedi e tanto pestato calli che avete raggiunto e superato la soglia della sopportazione. L'ordine dei commercialisti è composto da tecnici con i quali non vi siete mai confrontati alla faccia della concertazione e del rapporto con le categorie. Voi, infatti, avete aumentato tutti i redditi di tutte le fasce, di tutte le categorie economiche senza consultarne una.

significare perché con questa dichiarazione dei redditi non c'è impresa, non c'è cittadino e contribuente che non abbia visto aumentare il proprio contributo da dare allo Stato. Se questo è il cuneo fiscale, abbiamo capito dove lo abbiamo preso, caro Sottosegretario.

percorreremo quell'arduo e periglioso percorso della *probatio* *diabolica*». Voi, infatti, stabilite come noi cittadini dovremo giustificarci e su quali parametri perché nemmeno i libri contabili bastano; bisogna provare secondo i vostri criteri che non si è guadagnato. Loro, quindi, percorreranno questo percorso arduo e difficile e soprattutto lo consiglieranno come metodo a tutti i loro assistiti e clienti. Guardate che qua non siamo ancora alla rivolta fiscale, ma siamo fiscale, ma siamo appena dietro l'angolo. Questo Governo non può andare avanti in questa maniera. State propinando a tutto il Paese una cura da cavallo! Il guaio è che qua si sta rischiando che il cavallo non ce la faccia e non sopravviva. Pensateci un pochino!

prima di entrare nel merito della nostra discussione vorrei sottolineare un aspetto che credo sia rilevante per i lavori di questo Senato. Abbiamo oggi qui a rappresentare il Governo il sottosegretario Lettieri, a cui va il mio saluto e ringraziamento per essere presente, ma è certo che su una vicenda di questo genere il Senato avrebbe meritato la presenza del vice ministro Visco, il quale è responsabile di tutto questo. Mi rendo conto del fatto che il Vice ministro abbia qualche imbarazzo ad apparire in pubblico e, laddove si discuta del suo operato, forse avrebbe dovuto rispondere di più di una cosa;

sta abusivamente esercitando la delega che ha detto di aver rimesso o altrimenti sta esercitando una delega, che è stato detto esser stata rimessa in quest'Aula, ma non è vero che sia mai stata rimessa. Ricordo, signor Presidente, al Governo - e su questo vorrei una risposta in questo dibattito - che la legge prevede che la Guardia di finanza sia sotto la diretta responsabilità del Ministro e già alla nascita di questo Governo è stata compiuta una forzatura, attribuendo con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la delega al Vice ministro. Ciò detto, nel momento in cui ci è stato comunicato che il Vice ministro avrebbe rimesso le deleghe, non c'è stato atto di uguale forza giuridica dal quale risultasse a testimonianza del fatto che il Vice ministro o esercita legittimamente tale delega - e il Governo ha mentito in quest'Aula - oppure la esercita abusivamente. Resta il fatto che, non appena è stato nominato il nuovo comandante generale della Guardia di finanza,

incontro ufficiale, rendendo quindi omaggio al Vice ministro, a cui il Comandante generale della Guardia di finanza ritiene, in base ai fatti e alle norme, di dover rispondere. Su tale questione noi ci attendiamo una risposta

Ciò premesso, Presidente, oggi l'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni relative agli studi di settore. Capisco le semplificazioni del linguaggio che pongono la necessità di dare un oggetto chiaro e riconoscibile a tutti, tuttavia, non è questo l'oggetto della nostra discussione per una semplice ragione che cercherò di spiegare. E profitto del fatto che i nostri lavori vengono trasmessi in diretta radiofonica e televisiva per fornire qualche elemento di conoscenza anche ai cittadini che ci stessero ascoltando. Perché non stiamo parlando più, signor Presidente e colleghi, di studi di settore? Perché, secondo le definizioni ufficiali che leggo dal sito dell'Agenzia delle entrate e della SOSE (la società incaricata della gestione degli studi di settore), gli studi di settore sono il frutto di un accordo di reciproca collaborazione tra Amministrazione finanziaria, associazioni di categoria e ordini professionali. sono «lo strumento innovativo che consente un nuovo rapporto tra il fisco e il contribuente in termini di trasparenza, equità e certezza. sono uno strumento innovativo» - afferma l'Agenzia delle entrate - «in quanto si fondano sulla partecipazione e sulla condivisione da parte delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, basandosi su un sistema relazionale in cui Amministrazione finanziaria, contribuenti, associazioni di categoria e società per gli studi di settore, attraverso due strumenti, la commissione di esperti e gli osservatori provinciali, concordano gli studi». sono uno strumento meramente statistico con lo scopo, attraverso un regime concordato tra contribuenti e fisco, di dare un orientamento, ai fini delle valutazioni dei redditi di impresa, sia all'Amministrazione finanziaria, che riceve dagli ordini professionali delle categorie informazioni sull'attività economica nel territorio, sia ai contribuenti che ricevono dall'Amministrazione finanziaria livelli di consolidamento di questi dati e di formalizzazione sul piano non solo giuridico, ma anche su quello operativo, in modo tale che ciascuno sappia più o meno quanto la propria impresa

abbiamo una piena e totale condivisione. Anche nel periodo in cui abbiamo governato, abbiamo ritenuto di poterli potenziare in quel rapporto

rispetto alla realtà economica dei contribuenti; di adesione della realtà dei contribuenti rispetto agli elementi di valutazione dei redditi d'impresa e dei redditi professionali. Dal punto di vista giuridico e da quello operativo, il Governo, attraverso la legge finanziaria 2007, ha totalmente mandato in soffitta gli studi di settore e ha introdotto la catastizzazione del reddito e la *minimum tax* di fatto e di diritto. nella finanziaria, colleghi della maggioranza, che avete approvato con un voto di fiducia e che abbiamo cercato di combattere in tutti i modi, è stato dato un valore giuridico, la presunzione di validità legale - che non avevano - agli studi di settore. È chiaro che, se si deve difendere da uno strumento statistico in un rapporto di contraddittorio con il fisco, il contribuente deve avere degli spazi in cui poter dimostrare perché i redditi della sua impresa e i ricavi di quell'anno non sono coerenti e congrui con quello che lo studio presuppone. Se, però, dal punto di vista giuridico, lo studio assume una presunzione legale,

Questo stravolgimento giuridico dello studio di settore non ci consente di far altro che chiedere l'immediata sospensione degli indicatori di normalità - su tali indicatori interverrò dopo - - e ci porta a proporre l'abrogazione di quella norma della finanziaria per la quale lo studio di settore ha assunto valore di presunzione legale e quindi non è più studio settore com'era secondo la concezione per cui è stato introdotto e per la quale per cinque anni abbiamo lavorato, facendo crescere la base imponibile ed erodendo significativamente l'evasione fiscale. Ma c'è di più: lo studio di settore sia uno strumento concordato tra gli attori in gioco, che sono il fisco, da una parte, e le categorie produttive e gli ordini professionali, dall'altra, l'introduzione, attraverso la finanziaria prima e il decreto attuativo poi, ad opera di una sola parte - il fisco - degli indicatori di normalità economica. Essi non sono la manutenzione degli studi di settore, come ha detto il Ministro, ma un'altra cosa. Qualsiasi studente di economia sa benissimo che qualunque tipo di bilancio può essere interpretato attraverso indici, indici, che sono criteri di valutazione soggettivi e che possono avere finalità diverse. Voglio fare l'esempio di un imprenditore che conosco e che lavora, nel settore della pubblicità diretta attraverso i volantinaggi, per le società di grande distribuzione; la sua impresa ha contratti molto importanti in tutto il territorio nazionale con i principali gruppi della grande distribuzione alimentare. Egli ha provato ad approcciare anche altre imprese e, in un rapporto con la TIM, si è proposto come fornitore. Ebbene, la TIM, per le sue procedure interne, ha stabilito che il MOL (il margine operativo lordo) di quell'azienda non è adeguato alla sua griglia di valutazione e ha deciso di non affidarle lavoro. Questo discorso vale nella negoziazione tra i privati,

possibile fornitore o cliente e ne decide l'affidabilità. Ma inventare indici di normalità economica, introdurli per legge in uno strumento che diventa presunzione legale, è esattamente il modo attraverso il quale si può ottenere il risultato opposto allo studio di settore, cioè lo stabilire preventivamente quanto deve entrare. Tant'è vero che ciò è confortato dal fatto che abbiamo, sia che abbiamo, sia nella finanziaria che nel DPEF che l'ha preceduta, una previsione di incremento di gettito dovuto all'introduzione di indici di normalità economica. Invece, la la manutenzione degli studi di settore, in via di principio, non può prevedere incremento o decremento di gettito, perché essa, nel rapporto con le categorie e il mondo produttivo, fa sì che alcune attività in un certo periodo possano generare meno ricavi e meno profitti e altre possano migliorare. Quindi, non è presumibile stabilire *a priori* se la manutenzione degli studi di settore darà o meno incremento di gettito, tant' è vero che il Governo non ha scelto la strada della manutenzione, che aveva di fronte a sé, avendo tutti gli strumenti per farla e avendo la piena disponibilità di tutte le categorie produttive rappresentate nella commissione di esperti, nella SOSE e in ogni tavolo negoziale legato agli studi di settore; no, ha voluto utilizzare uno strumento arbitrario, è andato ad esaminare le simulazioni delle dichiarazioni degli anni in corso (è nelle dichiarazioni del vice ministro Visco, che poi voglio citare) e, sulla base di queste, si è accorto che le entrate erano insufficienti rispetto al fabbisogno che aveva deciso di introitare con gli studi di settore e ha posto i parametri di normalità economica non sulla base di fatti reali, ma dell'esigenza di cassa dello Stato. Questo ha portato Confesercenti e Confcommercio a dire che era ora che il Governo la smettesse di considerarli un Bancomat in cui venire a

Scusate, colleghi, ma credo che chiunque abbia vissuto in una realtà economica marginale (e spesso questo non capita, purtroppo, ai signori dell'Agenzia delle entrate o ai ai componenti del Governo in carica e dell'attuale maggioranza, che di altro hanno vissuto tutta la vita), chiunque abbia avuto un'impresa piccola, familiare, sa benissimo che quel reddito dichiarato alla fine è il reddito finale d'impresa depurato dal reddito individuale, che magari, come amministratori o prestatori d'opera, il titolare dell'impresa e i suoi familiari hanno già percepito durante l'anno, ed è sottoposto ad una tassazione IRPEF. Quel reddito d'impresa, una volta percepito dal titolare di impresa,

un gioielliere non possa guadagnare come un operaio: effettivamente non è così. Durante l'anno guadagna il compenso che ha deciso di attribuirsi e solo alla fine dell'esercizio ha un utile in più, su cui pagherà le tasse per il reddito d'impresa e le tasse sul reddito personale.

tra gli indicatori viene verificata anche la congruità tra gli ammortamenti portati in deduzione e il valore dei cespiti su cui l'ammortamento viene effettuato. Il Ministro, per gettar scandalo e per dire come i piccoli imprenditori, gli artigiani, siano una banda di evasori, ci racconta che 137 tassisti non hanno il taxi, pur avendone

a buon prezzo) ha sbagliato a non indicare il valore del suo mezzo, di cui ha messo una quota in deduzione. Questo cittadino va trattato come un evasore con un accertamento obbligatorio, o basterebbe una telefonata per dirgli che si è dimenticato di scrivere l'anno

così come cerca di mettere alla gogna 3.800 ristoranti che non avrebbero la cucina e tavoli di cui hanno dichiarato l'ammortamento: magari può capitare che l'ultima rata di ammortamento coincida con la dismissione

che per trent'anni sono stati costruiti per attaccarsi come sanguisughe alla giugulare del tessuto produttivo del Paese e ridurlo in condizioni di fiscalità impossibile.

perché tutti quelli che vengono sottoposti ad accertamento ordinario pagano almeno tre volte. Un messaggio del genere al mio paese si chiama avvertimento

sostenerla a chi nella maggioranza vede queste cose tra i propri elettori e nel Paese, perché solo sospendendo gli indicatori di normalità, questi strumenti di rapina, e ripristinando gli studi di settore invece che questa *minimum tax* e catastalizzazione del reddito con la presunzione legale potremo riprendere la strada di un'adesione tra il fisco e il contribuente. Altrimenti, la rivolta fiscale sarà benefica. *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso che la lotta all'evasione fiscale nel nostro Paese è un impegno necessario e meritevole di lode che, fortunatamente, sta già ottenendo dei risultati positivi, mi permetto di criticare la politica fiscale perseguita finora e in particolar modo l'applicazione degli studi di settore recentemente revisionati: essi non rappresentano assolutamente la realtà cui si riferiscono. Applicando i nuovi parametri degli studi di settore, emerge che un numero altissimo di imprese non è congruo. Soprattutto le medie, piccole e microimprese non riescono a rientrate nei parametri di congruità fissati dagli studi. Ed il motivo sta nel fatto che i nuovi indicatori di normalità economica non rispettano assolutamente la realtà economica del nostro Paese. Inoltre, mi preme sottolineare che trovo assurda ed inaccettabile l'applicazione retroattiva delle nuove regole degli studi di settore; un fatto unico in Europa! La certezza del diritto è un principio di civiltà giuridica che va assolutamente rispettato; la certezza dell'imposizione è di fondamentale importanza per i contribuenti. Gli studi di settore non possono, poi, essere uno strumento di accertamento fiscale automatico. Ribadisco il concetto che, così come revisionati, gli studi di settore siano inapplicabili e sbagliati. La mozione di maggioranza da me sottoscritta costituisce un primo passo nella direzione giusta; ma indubbiamente ne devono ne devono seguire altri. Come ho già ribadito più volte in quest'Aula, la politica fiscale e finanziaria del Governo ha bisogno di una svolta affinché l'economia italiana possa continuare a crescere; la nostra mozione è già - insisto - un buon inizio. Un punto importantissimo contenuto nella mozione, e da me più volte sollecitato, è la richiesta di abolire l'obbligo di presentazione dell'elenco clienti-fornitori. Per gli imprenditori quest'obbligo è visto come un mero aggravio burocratico privo di senso, e a nome loro chiedo al Governo la sua abolizione. Se la svolta nella politica fiscale e finanziaria, annunciata dal Governo, non verrà realizzata in tempi brevi, rischiamo fortemente che nelle zone di confine, ossia nel Nord d'Italia, moltissime imprese siano costrette a lasciare questo Paese per trasferirsi all'estero, cosa che già sta accadendo. Oltre a perdere le aziende e notevoli entrate fiscali, perdiamo soprattutto tantissimi posti di lavoro sicuri. Dobbiamo evitare che ciò avvenga. mi rivolgo nuovamente al Governo e chiedo un cambiamento, non a partire da domani, ma da oggi. È compito del Governo creare le condizioni giuste per favorire posti di lavoro sicuri e ciò non solo nel settore pubblico, ma soprattutto nel settore privato. I giovani che vogliono dar vita ad una impresa o succedere all'azienda familiare vanno incoraggiati e devono trovare un clima di fiducia. Trovo sia compito del Governo rimuovere tutti gli ostacoli, anche quelli burocratici, affinché un'azienda possa guardare con ottimismo al futuro. al futuro. Concludo dicendo che, dopo anni di stagnazione, questo Paese finalmente può tornare a crescere. Questa è una fase delicata ed è nostro compito dare al mondo imprenditoriale il necessario sostegno. Occorrono politiche di sviluppo e politiche attente soprattutto ai bisogni delle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale dell'Italia. L'economia sudtirolese, ma non solo, ha dimostrato in modo esemplare come le piccole e medie imprese possano crescere e diventare competitive a livello mondiale. Chiediamo, pertanto, al Governo di supportare le imprese nei loro sforzi e di sostenerle

*(SDSE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, non vi è dubbio che nel nostro Paese, nel nostro sistema produttivo ed economico, la presenza, il ruolo e la funzione delle piccole e medie imprese siano certamente rilevanti. Credo che queste vadano salvaguardate e debbano essere oggetto di attenzione e di politiche adeguate di sostegno. Il Governo Prodi in quest'anno di legislatura ha dedicato molta attenzione per rilanciare, con adeguate politiche, lo sviluppo e la competitività delle nostre imprese credo che in questo contesto un'attenzione particolare debba andare sempre più al sistema della piccola e media impresa, dell'artigianato e del lavoro autonomo. Accanto alle politiche di risanamento e di diminuzione della spesa pubblica, alle politiche di sviluppo, un elemento importante è stato ed è rappresentato da un'adeguata politica della finanza pubblica. In questo, un ruolo primario sta nella lotta per contrastare l'evasione fiscale, cercando di finalizzare questa battaglia al recupero di risorse da riutilizzare per ridurre progressivamente la pressione fiscale per le famiglie e le imprese, in particolare per quelle piccole degli artigiani e per il lavoro autonomo, per avviare nel contempo politiche in materia di lavoro attraverso un'efficace lotta al lavoro nero e precario e politiche di Stato sociale volte a favorire le fasce più deboli della popolazione. Ritengo che un'efficace e rigorosa lotta all'evasione fiscale sia uno dei presupposti essenziali per riportare equità nel rapporto fiscale e per fare in modo che non ci siano storture e concorrenza sleale nel mercato. mercato. Credo sia interesse di tutte le imprese che lavorano e operano correttamente farsi paladini e sostenitori di questa battaglia. Per tale ragione ritengo siano da combattere quei luoghi comuni, quelle affermazioni che vedono una automatica identificazione tra lavoro autonomo ed evasione fiscale, anche perché questi giudizi non trovano corrispondenza nei fatti e nei dati della realtà contributiva nazionale; credo altresì che non sia nemmeno accettabile un livello di evasione ed elusione fiscale ormai pari al per cento del prodotto interno lordo. Questi dati non sono sopportabili dal Paese e dallo stesso sistema di imprese perché ciò fa sì che il carico fiscale e tributario gravi tutto sull'economia legale, mentre le imprese che operano nel sommerso e nella illegalità possono operare a danno degli altri facendo una concorrenza sleale. Per questa ragione sarebbe necessario che le associazioni di rappresentanza e di categoria, oltre a far sentire la loro voce critica sull'eccessiva pressione fiscale (così come hanno fatto nelle assise, che si sono tenute in questi giorni, di artigiani e commercianti), dichiarassero e si impegnassero a dare un appoggio al Governo per la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale. In questo contesto credo che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e successivamente la finanziaria, abbiano fortemente innovato la modalità di accertamento dei redditi basata sugli studi di settore, che gli stessi rappresentino uno strumento di supporto alle attività di controllo e di accertamento e mettano in rilievo la necessità di una attenzione ai dati stessi che 1'Agenzia delle entrate utilizza come punto di riferimento, mettendo così in luce quelle situazioni di diversità o di disomogeneità da quei dati. Quindi, è bene ricordare e ribadire che gli studi di settore non sono fattore di accertamento automatico e dunque non sono nemmeno una *minimum tax*.

le revisioni devono essere realizzate attraverso un confronto vero e trasparente con le associazioni di categoria. Per questa ragione, noi crediamo che lo strumento degli studi di settore e il protocollo sottoscritto dal Governo con le associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, dell'artigianato e del lavoro autonomo rimangano uno strumento valido e che il loro valore si fondi sulla capacità di indirizzo e di comportamenti virtuosi dei contribuenti e che nell'accordo sottoscritto ci sia lo spirito di promuovere queste cose e porre il riequilibrio fiscale in misura proporzionale all'emersione della base imponibile. base imponibile. Ritengo di dover esprimere una perplessità sul metodo che si è seguito nell'elaborare i nuovi indici di «normalità economica» da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che si è discostato dal metodo concertativo: metodo e spirito che vanno decisamente recuperati,

anche i contenuti del comma 14 dell'articolo 1 della legge finanziaria, per ritornare invece ai contenuti del protocollo sottoscritto il 14 dicembre 2006, che prevede che gli «indicatori di normalità economica» debbano essere individuati con la partecipazione degli esperti delle categorie interessate, al fine di trovare indici «selettivi ed equi», in maniera da individuare comportamenti fiscalmente corretti. Per questo bisogna che vengano uniformati al protocollo anche gli indicatori di normalità economica, individuati con il decreto-legge del 20 marzo 2007, recuperando così un rapporto positivo con le categorie e ponendo le premesse per continuare insieme la battaglia all'evasione. Per questa ragione, ritengo ritengo importanti alcuni segnali arrivati dal Governo, quale, ad esempio, la decisione di prevedere il pagamento delle imposte entro il 1° luglio senza il pagamento della maggiorazione dello 0,40 per cento per coloro a cui si rendono applicabili gli studi di settore. Noi di Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo anticipiamo che abbiamo firmato e che sosterremo la mozione n. 114. Auspichiamo, quindi, che si continuino a valorizzare gli studi di settore, quale strumento di indirizzo e di armonizzazione del rapporto contribuente-fisco al fine di garantire principi di equità, certezza e trasparenza, a perseguire con convinzione il metodo concertativo per la revisione degli indici degli studi di settore, proseguendo nello spirito del protocollo del dicembre scorso, magari aggiornandolo e migliorandolo, che si tutelino il lavoro e i lavoratori, garantendo una ferma lotta al lavoro nero, e che si assicurino i diritti di tutti. Infine, crediamo che la lotta all'evasione e all'elusione debba rimanere uno degli obiettivi di questa maggioranza e di questo Governo.

avremo finalmente la risposta di Veltroni: siamo tutti in trepida attesa, perché non è come il Sottosegretario che è qui e che deve rispondere; ci sentiamo già tutti

la Baraldini e D'Elia sembra che stiano facendo pubblicità per pistole ad acqua., sono diventati buoni. Persino Marino, il presidente della Commissione sanità, che si sta occupando della «dolce morte», sta pensando che prima di fare l'iniezione finale daremo un bel bacino. Quindi, onorevole Sottosegretario, non la invidio; tutti stiamo aspettando questo. Ma c'è l'altro psicodramma: quello del tesoretto. Gli italiani non sanno più cosa succede perché quella del tesoretto è una favola bellissima e infinita. Vede, Presidente,

Alice nel Paese delle meraviglie, vi è la sorpresa di Padoa-Schioppa: un miliardo in più nel tesoretto.

Le dichiarazioni si spendono e questo fa il pari con tutte le altre: il tesoretto è di 2,5 miliardi di euro il 19 giugno; il 21 giugno sale già un po' meno, ma il 25 giugno è a 3,5 miliardi; i conti pubblici sono risanati l'8 maggio, ma il 22 giugno invece non sono più risanati e vanno ancora male. Tutti i giorni diamo i numeri, ma li diamo perché siamo furbetti; i furbetti ci sono e non sono solo quelli delle telefonate, i cattivoni che avevano le banche, ma sono

maggio, era cresciuto del 16,3 per cento e quello prodotto dall'IVA del 13,6 per cento; a settembre, poi, quando i tecnici del Governo si sono seduti, nei primi sette mesi dell'anno hanno registrato un 12,6, a fronte di un 9,4. Quindi, nel primo trimestre c'è stata una maggior crescita e c'è da dire che, da quando è arrivato il Governo Prodi - devo contrastare i dati che sono stati citati - la crescita è stata minima

non si voleva dare il merito a Silvio Berlusconi. Per carità! Diamo piuttosto il merito alla paura che gli italiani avevano nel veder arrivare finalmente il Governo del rigore.

dei conti non in ordine, del buco - oh mamma mia! C'era il buco - si è calata la mazzata fiscale sulle teste dei contribuenti: una manovra da 35 miliardi, composta per il 70 per cento da nuove entrate, con una pressione fiscale salita al 47,7 per cento. E poi qui arriva il tesoretto. Che bello, il tesoretto! Chissà dove lo vorrà mettere Veltroni! Darà tutto a tutti. Moltiplicherà i pani e i pesci: c'è già riuscito qualcuno, ma sono convinto che lui sicuramente saprà fare meglio. alla redistribuzione del tesoretto, mi fa piacere ricordare le tante promesse. Il presidente Morando giustamente diceva che è sbagliato spendere il tesoretto per lo scalone la spesa sociale italiana è gravemente squilibrata a favore della componente previdenziale. Giustamente egli parla di giovani, parla di bambini e dice che non si può mettere a carico dei più poveri e dei più giovani la più iniqua delle imposizioni fiscali. Mi sentirei di sottoscrivere questo. Non si può mettere a carico della fiscalità generale la spesa previdenziale, e questo è stato già fatto. Vorrei però ricordare al Presidente che il tesoretto è già andato dappertutto, magicamente ha già sanato l'ICI. Peccato che dai conti fatti dalla Confedelizia l'ICI si triplica; poi, arriva Rutelli e anche lui l'abbatte. Ma non basta dirlo sui giornali. Gli italiani vogliono vederlo nel proprio portafoglio. Vi lamentavate che Berlusconi annunciava. Caspita: Berlusconi è un dilettante nel fare annunci.

che dalle prese di posizione del Governo la parola famiglia è completamente sparita. Certo, è arrivata la nota dei teodem

che ha giustamente suscitato la contrarietà di tutto il mondo delle associazioni, anche perché gli indicatori sono stati determinati unilateralmente, sono fuori del contesto metodologico degli studi, retroagiscono all'anno 2005 in deroga allo Statuto dei contribuenti. Questo, dunque, è un segnale estremamente negativo di come la certezza del diritto vada a finire in soffitta, lì dove

Signor Presidente, onorevole sottosegretario Lettieri, non vorrei che questo dibattito fosse un'anticipazione del DPEF, anche per le cose dette dall'onorevole Polledri, e soprattutto non auspico un «modello Veltroni», che è fatto, ad esempio, di poca ICI in meno e di tanta addizionale IRPEF in più. Questo per chiarirci subito le idee. Oggi, per iniziativa dell'opposizione, è posto all'attenzione del Parlamento il problema degli studi di settore. Una questione che, come UDC, avevamo costantemente richiamato in ogni occasione parlamentare: nella finanziaria 2007, nei ripetuti interventi correttivi dei decreti Bersani-Visco, sul provvedimento *desaparecido* sugli ammortamenti per i beni immobili e per l'IVA auto e, più recentemente, sull'atto di indirizzo per gli obiettivi triennali di politica fiscale. Avevamo posto l'esigenza di intervenire rispetto a scelte dissennate operate da questo Governo. Ma il Governo è rimasto sordo agli appelli, un po' tardivi, anche della sua maggioranza e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Avevamo sottolineato con forza l'assurdità di quelle scelte era di tutta evidenza che il vice ministro Visco aveva imboccato una strada sbagliata e pericolosa. Quanto sta accadendo è la chiara dimostrazione della distanza abissale, incolmabile tra questo Governo e il mondo delle imprese. C'è una prima questione: il Governo, che proclama il metodo della concertazione, ne ha travolto ogni significato con un'interpretazione unilaterale rispetto al protocollo d'intesa del 14 dicembre scorso, ripudiando tale criterio, senza alcun coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'approfondimento e nell'elaborazione del sistema di accertamento diretto.

prescindendo quindi dalle risultanze delle scritture contabili cui sono tenuti i soggetti di imposta che esercitano attività di impresa o libero-professionale.

I limiti obiettivi degli studi di settore sono stati nel tempo ritenuti inadeguati in relazione all'impossibilità di poter predeterminare concreti parametri reddituali, che corrispondano alle obiettive realizzazioni del reddito, in relazione a varianti che attengono al settore di attività e all'ubicazione geografica dell'azienda e anche all'ammontare del PIL della zona geografica in cui opera il contribuente. È proprio per questi motivi che gli accertamenti basati sugli studi di settore non hanno avuto ampia applicazione, tenuto conto del constatato negativo impatto che accertamenti del genere hanno avuto davanti ai giudici tributari, che hanno in gran parte annullato gli atti di accertamento degli uffici basati su tali indici. Il professor Visco, tornato da vice ministro alla direzione della politica fiscale, si è affrettato tra l'altro a rivitalizzare gli studi di settore per farne un oppressivo strumento nei confronti dei contribuenti lavoratori autonomi, e parte la generale critica di fondo che riguarda la proposta di applicare anche ai redditi dichiarati nello scorso 2006 i parametri degli studi di settore determinati nel 2007, disattendendo platealmente i criteri generali dello statuto del contribuente, che sancisce l'irretroattività delle disposizioni tributarie. Inoltre, tali studi sono stati predisposti senza alcuna intesa o collaborazione con le associazioni di categoria. Ma è lo stesso professor Visco a dare la misura dell'inattendibilità degli studi di settore predisposti per il 2007 quando il suo stesso ufficio studi fa sapere che solo il 53,8 per cento dei lavoratori autonomi è entro i limiti dei criteri previsti di redditi presuntivi. È ben evidente che quando si è di fronte a tali macroscopiche differenze non si può agire con la minaccia degli accertamenti, che, di fatto, sarebbero impossibili. Infatti, si tratterebbe di verificare più di tre milioni di contribuenti a fronte di una capacità operativa di tutta l'Amministrazione finanziaria (civile e militare) che non supera la soglia dei 100.000 controlli sostanziali annui. Siamo di fronte ad un caso di grida manzoniana e questo il professor Visco lo sa, perché diversamente avremmo non il paventato sciopero fiscale, di cui qualcuno imprudentemente ha parlato, ma una giusta e civile disobbedienza civile da parte di quei cittadini che non possono essere chiamati a pagare imposte che non rappresentano la realtà reddituale di ogni singolo contribuente, in ossequio all'articolo 53 della Costituzione. Di questo però non c'è traccia nella lezioncina del professor Cipolletta, che si dedica alla politica economica più di quanto non faccia per illuminare il Paese verso un miglioramento della efficienza del trasporto ferroviario italiano, di cui ha assunto la responsabilità attraverso una decisione di questo Governo. Gli indicatori sono stati stabiliti in maniera frettolosa, approssimativa, direi rozza. Questa vicenda fa il paio con quanto accaduto con il catasto terreni, dove sono stati registrati clamorosi errori che hanno comportato anomalie grossolane nella classificazione della qualità delle colture. Voi, in base a quel modello, state procedendo alla catastizzazione dei ricavi! Volete utilizzare uno strumento «di massa» che non è in grado di rappresentare in modo compiuto l'attività economica di ogni singolo contribuente, perché non tiene conto di elementi contingenti relativi all'ubicazione dell'impresa e alla validità del contesto economico e sociale. Anziché individuare strumenti veramente selettivi di equità fiscale, che richiederebbero un forte impegno nel contrasto della concorrenza sleale, nella contraffazione, nel lavoro sommerso e nell'evasione fiscale,

mentre da parte nostra sarebbe auspicabile una riforma di grande impatto sui comportamenti dei contribuenti, che affermi in modo esplicito il principio del contrasto di interesse tra i vari soggetti di imposta. Ma come si fa a sostenere che tale principio è una «balla colossale», come ha affermato il vice ministro Visco, che evidentemente è fuori dalla realtà? La lotta all'evasione deve essere condotta nel rispetto dei principi di civiltà giuridica e fiscale. Come si fa a inserire questo meccanismo posticcio, mutuato da esperienze straniere, senza una revisione radicale dell'intero sistema, in grado di recepire quei meccanismi nell'ambito di un'architettura fiscale coerente e organica? Una vera razionalizzazione del sistema e una sua semplificazione passano non attraverso l'inasprimento fiscale, che ha finito per colpire i contribuenti onesti, ma attraverso un'attività di accertamento più efficace. Il sistema italiano è ben diverso; in altri sistemi il conflitto di interesse tra cittadini e fisco viene risolto attraverso un ampio riconoscimento della deducibilità delle spese dal reddito disponibile. L'introduzione del conflitto di interesse diviene base di solidarietà fiscale, andando nella direzione opposta a quella praticata da Visco, dunque, non al restringimento di spese fiscalmente deducibili, ma a favore di un più generoso riconoscimento di queste ultime. Anche nei giorni scorsi il Ministro dell'economia e delle finanze, alla festa nazionale del Corpo della Guardia di finanza, si è lasciato andare a giudizi demagogici. Non prende atto di avere prodotto provvedimenti legislativi sbagliati, in una confusione normativa e in un contesto di politica fiscale che hanno avuto negative ripercussioni sui sistema delle piccole e medie imprese, di quelle artigiane e di quelle commerciali, che hanno visto aggravarsi non solo i conti fiscali veri e propri ma i costi di gestione del sistema tributario di impresa. Ha voluto presentare una società dei contribuenti italiani come evasori, trasformandoli in intermediari e ausiliari del fisco. Come non vedere i rischi che la nuova disciplina produce, tra cui un aumento delle attività di verifica per effetto degli indici di coerenza e di normalità economica introdotti, che appaiono eccessivamente oscillanti? Volete dare validità a ciò che non è valido perché la maggior parte delle piccole e medie imprese sta fuori dai paramenti stabiliti unilateralmente e che sono privi di validità statistica. Vi è poi un'altra questione di straordinario rilievo: la violazione di princìpi fondamentali relativi alla irretroattività delle norme fiscali, che stanno alla base dello statuto per il contribuente. Mi domando se il Governo abbia letto attentamente la relazione della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, appena trasmessa alla Commissione finanze; se abbia letto accuratamente le relazioni del Garante per il contribuente, figura istituita in tutte le Regioni d'Italia; se abbia visto le violazioni che riguardano appunto l'eccessiva pressione legislativa sia nei livelli, in nuovi e pesanti adempimenti, sia nell'applicazione retroattiva delle disposizioni. Questi nuovi studi di settore rischiano di innescare accertamenti o presunzioni di colpevolezza che rievocano la *minimum tax*. Sono appunto una *minimum tax* mascherata. L'imposta minima, infatti, prescinde dal principio della tassazione del reddito prodotto per rifarsi al concetto di reddito "normale", stabilito dall'Amministrazione finanziaria. Si realizza così un sistema di imposizione di reddito normale, che consentirebbe un appiattimento per i soggetti che si trovassero oltre la soglia minima richiesta. Vi è l'abbandono del principio di accertamento basato sulle scritture contabili obbligatorie, una rottura rispetto ai princìpi di contabilità, una lesione dei princìpi costituzionali, in quanto rappresenterebbe una deroga rispetto alla tassazione del reddito prodotto e un riconoscimento all'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti. Occorre ripristinare il valore probatorio della contabilità ordinaria, che non viene rispettato. Ecco perché vogliamo una moratoria. Vogliamo il ripristino del metodo della concertazione. Vogliamo che si ritorni al protocollo di intesa di dicembre. Si elimini la retroattività per il 2006, si ritorni al valore sperimentale degli studi di settore, si ripristini un clima di fiducia tra fisco e contribuente, tra Amministrazione finanziaria e categorie. Le inefficienze dell'amministrazione non possono essere scaricate né sulle categorie produttive né sulle categorie professionali. Avete cambiato le regole del gioco a partita in corso. Vogliamo una revisione complessiva del sistema che realizzi un'autentica semplificazione fiscale, indispensabile per creare un nuovo clima di solidarietà, perché voi state mortificando le imprese e comprimete le possibilità di crescita e di sviluppo economico. Avete rinunciato a governare e a ridurre la spesa pubblica e compensate queste vostre incapacità aumentando la tassazione dell'impresa produttiva. Avete preferito minacciare piuttosto che avanzare proposte serie ed efficaci, come l'esclusione, per esempio, per le imprese che lavorano in conto terzi visto che sono nell'impossibilità di sottrarsi al fisco. Nella mozione di maggioranza vi è solo una difesa pasticciata dell'azione di Governo; sono evidenti tutte le contraddizioni della coalizione, l'incapacità di formulare proposte serie; vi muovete dentro regole che non sono né certe né eque. Vi è mancato il coraggio di affrontare la questione per il verso giusto, che era quello, per esempio, del *change over* dell'euro. Quella era la strada per affrontare lo spostamento di ricchezza, ma non ne avete avuto il coraggio perché si sarebbe risalito alle vostre pesanti responsabilità sul valore del concambio. Vi è soprattutto la contraddizione tra statuto del contribuente e efficacia retroattativa degli studi di settore che non viene rimossa. Non vorremmo, Presidente, che alla fine di tutto questo disattento dibattito, rispetto a una questione invece importante, l'unico beneficiario di questa mozione fosse ancora una volta il Trentino Alto Adige con i riferimenti non alle aree marginali del Paese, ma al voto marginale del Senato. Questa vicenda degli studi di settore è il fallimento della politica fiscale del Governo. Presidente, voglio sottolineare soltanto una cosa. In quel provvedimento *desaparecido*, cui facevo riferimento prima, c'era un ordine del giorno della stessa maggioranza o di parti della maggioranza (quella che scrive le lettere sui giornali perché non ha il coraggio di assumere posizioni concrete in quest'Aula) in cui si chiedevano cose certamente diverse. Si diceva, per esempio, di riaprire immediatamente il dialogo costruttivo con le categorie economiche, di stabilire che gli indici di normalità economica introdotti con gli studi di settore non fossero applicabili all'esercizio 2006 e avessero valore sperimentale. Queste sono le cose che scrivono su un documento rispetto ad altre cose che invece vengono poi prese in esame nella mozione Questa è la contraddizione. Non vorrei che invece di andare verso il partito democratico si andasse verso la doppiezza togliattiano. Presidente, concludo questo mio intervento rappresentando solo degli auspici, perché non mi faccio illusioni rispetto alla capacità di questa maggioranza di affrontare e realizzare obiettivi seri di politica tributaria e di lotta all'evasione, che passano però e soprattutto attraverso un nuovo Governo e un nuovo Ministro dell'economia e delle finanze.